Signor Presidente, innanzi tutto le auguriamo un buon giorno. Vorrei semplicemente reiterare la richiesta, a nostro giudizio positiva, del presidente Calderoli, il quale giustamente riteneva opportuna,

quindi seguito alla procedura avviata con decreto, che però giace ancora presso la Corte dei conti. Vorrei ricordare ai colleghi e a lei, Presidente, che senza registrazione della Corte dei conti il decreto non è efficace.

studiate, analizzate e approfondite e che poi ci sia un esito favorevole che possa sbloccare la procedura e portare alla registrazione del decreto. ci fosse l'insediamento del Comandante generale questa mattina o comunque prima della formalizzazione della registrazione del decreto, tale insediamento sarebbe assolutamente invalido e illegittimo e creeremmo un caos istituzionale che non ha precedenti nella storia del Paese. Vogliamo anche ricordare, signor Presidente, a futura memoria

a discutere è inteso a definire un nuovo assetto complessivo della disciplina di un settore particolarmente delicato e che purtroppo ancora oggi occupa

diverso non tanto per i contenuti della delega, che peraltro sono stati puntualizzati ed ulteriormente articolati, quanto per la scelta, da tutti i Gruppi e sostenuta anche dal rappresentante del Governo, di introdurre, accanto alla disciplina di delega, un insieme di disposizioni immediatamente precettive contenute negli articoli da 2 a 11 -, in considerazione del carattere di urgenza e di drammaticità che presenta il problema della sicurezza sul lavoro. una grave piaga sociale che gli articoli da 2 a 11 del provvedimento intendono affrontare da un lato con il potenziamento e con un maggiore coordinamento dell'attività di vigilanza e dall'altro con misure per rafforzare l'azione di prevenzione. Nell'elaborazione dei predetti articoli la Commissione ha tenuto presenti anche i contenuti del disegno di legge n. 1486, di iniziativa del senatore Sacconi ed altri, il cui esame si è svolto congiuntamente con il disegno di legge n. 1507; inoltre, ha largamente attinto dall'approfondito lavoro di elaborazione e proposta svolto sia nella passata che nell'attuale legislatura dalla Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro, il cui contributo ha anticipato alcuni contenuti del disegno di legge in esame. Ai fini della predisposizione del testo sono state altresì utili le audizioni informali svolte presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione. Infine, il dibattito in Commissione ha evidenziato che una politica più incisiva di tutela della sicurezza sul lavoro non può prescindere da un impegno conseguente anche sul piano della spesa.

poiché nei successivi articoli sono contemplate disposizioni onerose, ad esempio l'assunzione del personale ispettivo ed il credito d'imposta per una quota delle spese di formazione per la sicurezza sostenute dal datore di lavoro. In conclusione, è doveroso da parte del relatore esprimere un vivo ringraziamento ai rappresentanti del Governo che hanno preso parte al dibattito e manifestare un vivo compiacimento per l'elevato livello di discussione in Commissione, che si è svolta in un clima di collaborazione dialettica tra i Gruppi di maggioranza e di opposizione, i quali, pur nella distinzione delle posizioni politiche, hanno profuso un comune impegno per dare vita ad un testo quanto più possibile condiviso, cercando così di recepire nel metodo di lavoro oltre che nei contenuti il significato dei moniti più volte rivolti dal Capo dello Stato sui temi della sicurezza

Presidente, prendo la parola per confermare un annuncio che informalmente avevamo già fatto pervenire agli uffici della Presidenza

che pensiamo più utilmente di far esaminare dall'Aula attraverso gli emendamenti che l'*iter* del provvedimento. Invero, noi siamo convinti che quei dubbi relativi alla stessa costituzionalità del disegno di legge e che riguardino in modo particolare la corretta applicazione dell'articolo 117 della Carta costituzionale, laddove stabilisce in modo inequivoco una competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di sicurezza del lavoro, interpretazione che è stata oggetto di due pareri del Consiglio di Stato in occasione dell'esame trascorsa legislatura di un analogo provvedimento e del conseguente decreto delegato. In quella sede il Consiglio di Stato, in modo particolare, ebbe a sottolineare come il provvedimento di legge dovesse limitarsi a declinare i princìpi fondamentali e a indicarli esplicitamente, in modo che il legislatore regionale potesse poi operare all'interno di essi con il dettaglio necessario. Analogamente, avevamo presentato un'eccezione di costituzionalità riferita alla alla mancanza di copertura di un provvedimento che complessivamente rafforza i doveri del datore di lavoro, ricordandoci che il datore di lavoro è anche la pubblica amministrazione con gli oneri che conseguentemente si determinano. proposte sottolineo anche quella relativa ad un impianto sanzionatorio che ci appare non corrispondere ai criteri costituzionali che vogliono una proporzionalità adeguata tra la la sanzione e la violazione per la quale essa viene disposta. Infine, ricordo la considerazione relativa alla indeterminatezza dell'oggetto, come si riscontra spesso nelle deleghe: deleghe che possono definirsi talora in bianco, sottraendo al Parlamento la propria essenziale funzione.

e ciò è avvenuto nonostante i dissensi che in quella sede si sono manifestati e che, sempre in Commissione, non sono stati sanati, tanto che quegli emendamenti sono stati riproposti in una misura assolutamente compatibile con un rapido esame del provvedimento. Quindi, concludendo, è a quegli emendamenti che voglio fare riferimento; sarà quella la sede nella quale quegli stessi contenuti saranno esaminati nell'obiettivo di perseguire obiettivamente risultati migliori in termini di salute e sicurezza nel lavoro perché è dei risultati che ci deve interessare. Troppo spesso l'approccio appare formalistico l'approccio appare formalistico e ricordo che soprattutto nelle dimensioni di impresa, nei settori più esposti alle minacce che si determinano nei confronti della salute e della sicurezza del lavoratore, soprattutto in quegli ambiti del nostro tessuto produttivo, il tradizionale impianto regolatorio e il tradizionale impianto sanzionatorio si sono rivelati ineffettivi. Tale ineffettività si riscontra ancora nell'impianto di questo provvedimento.

che il Governo intende far svolgere la cerimonia della presa dei poteri del nuovo Comandante generale della Guardia di finanza. Mi pare che questo sia un atto indebito e illegittimo e che costituisca una evidente intimidazione. La Corte dei conti non ha registrato il decreto. Sollevai questo problema in Aula dicendo che sarebbe stato opportuno svolgere un dibattito dopo aver avuto notizie della registrazione del decreto e mi fu risposto che non era un fatto rilevante e che esistevano addirittura delle indiscrezioni secondo cui il decreto sarebbe stato registrato senza difficoltà. Oggi apprendiamo che le mie preoccupazioni erano perfettamente giustificate,

Tutto questo proviene da un Governo fortemente, chiaramente discreditato, indebolito, privo di autorevolezza davanti alla pubblica opinione, che sostituisce con la prepotenza la mancanza di autentica autorevolezza. Credo che il Senato debba intervenire su una questione che tocca princìpi fondamentali e non di cortesia istituzionale, ma di correttezza nella gestione delle istituzioni.

che riguarda i poteri dello Stato e chi il potere non ce l'ha ancora e non gli è stato attribuito perché ancora non è stato percorso l'intero *iter* rispetto al quale il giudice della possibilità di verificare la titolarità di un rapporto non si è ancora pronunciato. Fare oggi quello che si ritiene di fare è un oltraggio alla Corte dei conti ed è una mancanza di riguardo a ciò che rappresenta la separazione dei poteri, quello giurisdizionale che attiene alla Corte dei conti nella fase in cui ha il compito di verificare la regolarità degli atti. Quello che sta facendo il Governo è grave e non possiamo farlo passare in ragione o uno nemico. I Governi devono svolgere la loro funzione nei confronti della realtà del Paese, che è rappresentato da tutti noi qui dentro. Non è lecito che si possa consentire a chi ancora non ha titolo per farlo di esercitare una funzione per cui non è titolato; è grave che il Governo faccia questo. Non voglio entrare nella polemica se il Governo è prepotente perché è debole oppure perché la prepotenza fa parte di un tipo di interpretazione del proprio ruolo. Rilevo che oggi la Corte dei conti ha chiesto notizie - e le ha avute - e deve ancora decidere. Prima che si decida non è possibile che si svolga un ruolo di cui il soggetto non è titolare, chiunque sia. È molto grave questo. Mi dispiace. Sono un vecchio parlamentare, ma non ho mai visto queste cose prima di questa alba tragica della democrazia italiana.

quando l'atto non è ancora perfetto, e in assenza della registrazione della Corte dei conti non è ancora legittima, per così dire, l'acquisizione dell'incarico,

gran parte della materia dovrebbe essere di competenza regionale, mentre il provvedimento, così come impostato, salta completamente questo passaggio.

una legge delega che lascia al Governo ampia facoltà di intervento, con tempi assolutamente non certi (addirittura, se sommiamo tutte le possibilità, andiamo in là di anni per giungere al provvedimento

fa le cose in regola e le leggi già le rispetta mentre lascia completamente fuori, prima e dopo, chi vive e lavora in clandestinità), ci sembra veramente il modo e l'atteggiamento mentale più sbagliato. Ciò non di meno,

*(FI)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, i provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie impongono il riassetto*...

Come dicevo, i provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie impongono il riassetto della materia in oggetto, nel rispetto dell'equilibrio tra Stato e Regioni, per garantire l'uniformità della tutela della salute dei lavoratori sull'intero territorio nazionale. È dunque condivisibile lo sforzo di riordinare, coordinare, armonizzare e semplificare le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, prodotto dal legislatore nell'articolato in discussione,

cito alcuni: il mancato coordinamento dei provvedimenti che investono la molteplicità delle attribuzioni dei Ministeri, la mancata collegialità nella definizione dell'azione normativa del Governo, stanti le diverse e complesse competenze in materia; la mancanza di chiarezza sulle attribuzioni alle Regioni, e nello specifico in materia di monitoraggio, controllo e verifica, relativamente alle modalità dell'organizzazione del sistema di partecipazione e concertazione e gestione della formazione e informazione; la non individuazione di criteri e vincoli certi per la predisposizione delle linee guida (ad esempio principio di sussidiarietà, ruolo delle agenzie, della Conferenza delle Regioni e delle società scientifiche). In particolare, anche il riordino della materia stessa, la mancanza di estensione del campo di applicazione, anche quello che è al di fuori del rapporto di lavoro subordinato, gli obblighi espliciti per i preposti, così come menzionato nell'articolo 8, l'allargamento della platea della tutela e delle nuove forme contrattuali previste dal decreto legislativo 10 dicembre 2003, n. 276, nonché alle imprese familiari e ai lavoratori autonomi, così come già aveva previsto la legge Biagi; il mancato recepimento di alcune importanti direttive europee, come quella sull'amianto, sul rumore, sugli agenti fisici, in particolare le vibrazioni. Vi sono poi altri punti critici. Parliamo, ad esempio, dei lavori atipici. Per il lavoro a progetto si pongono tutele inferiori rispetto a quelle previste dall'articolo 66,

Per il datore di lavoro vi sono minori responsabilità. Non è, ad esempio, riportato l'attuale articolo 1, comma 4, della legge Biagi, dove sono stabiliti gli obblighi del datore di lavoro o dei dirigenti, il che farebbe venir meno, comunque, l'obbligo di controllo da parte del datore di lavoro sull'operato del suo stesso dirigente, l'obbligo nell'affidare i compiti di tener conto, oltre che delle capacità, anche delle condizioni soggettive degli stessi; l'esercizio del controllo circa l'operato del medico competente - sottolineo competente (articolo 4, comma 5) - e l'obbligo di custodia della cartella sanitaria e di rischio. sono poi norme di buona tecnica e di buona prassi. Il testo unico prevede il passaggio da una gestione della sicurezza per regole ad una per obiettivi. Quindi, assumono grande importanza norme di buona tecnica e prassi, anche se va chiarito il rapporto tra le norme abrogate e quelle dichiarate come di buona tecnica dall'articolo 5. Occorre dunque inserire una serie di nuovi elementi in aggiunta a quelli previsti, nei quali l'attuazione di quanto sopra richiamato sia espressamente rimandata alla predisposizione di apposite linee guida per l'applicazione della buona prassi della buona tecnica, all'individuazione dei criteri di certificazione delle stesse e all'individuazione dei soggetti incaricati di certificare e verificare il rispetto delle linee guida.

con una chiara, seppure indiretta, depenalizzazione, essendo su di esse previsto solo un potere di disposizione degli organi di vigilanza. Va richiamata poi la diversità tra lenorme di buona tecnica, in genere molto precise, e quelle di buona prassi, che derivano da comportamenti condivisi. Fino alla conclusione di questo processo dobbiamo mantenere viva la normativa esistente. Va chiarito l'ambito, sicuramente tecnico, dell'elaborazione, mentre per le norme attuative appare più funzionale attribuire alle Regioni un'esclusiva competenza in materia. La bilateralità e la valorizzazione del contributo delle forze sociali rappresentano un altro punto importantissimo. Gli organismi paritetici sono difatti i depositari della formazione. Determinante ed importante è il ruolo che potranno avere gli organismi bilaterali, per i quali va precisato rigorosamente il livello: regionale, provinciale, di distretto produttivo, subprovinciale, di settore e di comparto. Il testo unico sottolinea la necessità di valorizzare adeguatamente il dialogo sociale sul territorio e la bilateralità quale fattore determinante di controllo sociale, inducendo così le imprese a perseguire condotte socialmente responsabili. Presidente, il testo unico contrae la platea degli attori negli organismi di competenza istituzionale; non raccoglie le disponibilità di alta professionalizzazione maturate in questi anni e protagoniste nel campo della sensibilizzazione delle informazioni e della formazione e non coglie tutte le potenzialità che la società italiana può mettere a disposizione nell'ambito della ricerca, della consulenza e soprattutto dell'assistenza. Nelle relazioni sindacali promuove la bilateralità, ma rappresenta la riunione periodica come un semplice adempimento formale piuttosto che come un indispensabile strumento di comunicazione, informazione ed arricchimento delle reciprocità. alcuni princìpi preventivi. Si reintroduce il principio della massima sicurezza concretamente attuabile, principio superato da quello della massima sicurezza tecnicamente possibile.

la cui portata appare solamente limitata alla mera individuazione delle misure preventive e protettive. Scompare così l'autocertificazione, ma il documento può essere redatto in forma semplificata sulla base di indicazioni fornite dagli organismi paritetici. La previsione non è di per sé criticabile se non per il fatto che estende tale possibilità alle aziende fino a 50 dipendenti. Ciò svuota di significato il documento di valutazione dei rischi. Vorrei parlare anche di sorveglianza sanitaria, signor Presidente. Nella sorveglianza sanitaria non emerge la consapevolezza che il sistematico coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze in azienda, nell'organizzazione del lavoro, nei tempi e nella qualità del lavoro, nella gestione delle emergenze e dei rischi rappresenta un'importante fonte di indicazioni procedurali, accorgimenti comportamentali, sottolineature operative, fondamentale per raggiungere l'ambizioso obiettivo di sostituire un sistema per regole con uno per obiettivi. La sorveglianza sanitaria appare avere un ambito più limitato dell'attuale, estendendosi nei casi previsti dal presente decreto legislativo all'articolo 23, comma 1, e non alla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 16. Dovrebbero essere previste modalità di sorveglianza sanitaria ed adempimenti relativi (tenuta di cartelle sanitarie e di rischio, consegna, invio all'ISPESL) specifiche per i lavoratori atipici in particolare, tenuto conto delle peculiarità organizzative e temporali di tale attività; ad esempio, dovrebbe essere prevista una procedura più snella e realisticamente percorribile per la visita preventiva dei lavoratori interinali. Vorrei parlare infine del medico competente, signor Presidente. I requisiti delle altre figure professionali sono di alto livello, compresi i corsi di formazione specifici, mentre con la definizione di medico competente attualmente riportata nel testo unico viene invece sacrificata la professionalità del medico stesso. Non è stato modificato il ruolo del medico competente nel processo della valutazione del rischio; il medico competente deve partecipare attivamente e responsabilmente alla valutazione del rischio, sin dal suo inizio.

1.226, 1.10, 1.232, 1.233, 1.105, 1.0.201, 1.0.4, 1.0.206, 1.0.207, 2.202, 2.203, 2.204, 5.0.200 e 8.200. il disegno di legge all'esame dell'Aula conferisce, in sostanza, una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La strada del testo unico è una strada intorno alla quale si lavora da più anni, da più di un decennio, ed è una strada per noi condivisibile. A questo proposito, vorrei ricordare che nella passata legislatura, su delega conferita al Governo con l'articolo 3 della legge n. 229 del 2003, fu varato, attraverso lo strumento del decreto legislativo, il testo unico in materia di norme sulla sicurezza del lavoro; decreto successivamente ritirato, soprattutto a causa dei rilievi mossi presso altre sedi istituzionali circa la presunta violazione delle norme costituzionali in materia di riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni. L'attuale Governo sembra avere più fortuna con le Regioni. Ce lo auguriamo, perché, per un'effettiva applicabilità delle norme in materia di sicurezza, abbiamo bisogno di una legislazione snella e chiara. Non è più rinviabile, pertanto, l'operazione di procedere ad una semplificazione di un sistema normativo che raccoglie provvedimenti datati, rivenienti dagli ultimi cinquant'anni, ed improntati, fra l'altro, a princìpi di logica giuridica differenti rispetto all'impianto comunitario. Semplificazione, quindi, accompagnata da una revisione di numerosi profili, attesa l'evoluzione che ha interessato e interessa il mondo del lavoro. Il Gruppo di Forza Italia in Commissione si è astenuto e ciò nonostante l'ottimo lavoro, che qui va richiamato, svolto dalla Commissione nella sua interezza; astensione, dunque, nonostante più di qualche positività presente nel disegno di legge. Senza richiamare l'estensione della norma a tutti i settori, che costituisce per noi un aspetto condivisibile, perché nel passato l'applicazione della legge n. 626 del 1994 ha conosciuto deroghe di vario tipo, specialmente per la pubblica amministrazione, con l'aspetto positivo, e con altri particolarmente significativi, afferente l'inserimento della materia della salute e sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici e universitari e nei percorsi di formazione, finalizzata alla sensibilizzazione e alla informazione dei giovani. Tale scelta, infatti, si pone in linea con i più recenti orientamenti comunitari, ove l'insegnamento della materia della salute e sicurezza sul lavoro nelle politiche educative è uno degli obiettivi inseriti nel 6° Programma quadro comunitario, programma che ha fra le sue finalità quelle di formare giovani lavoratori che, una volta entrati nel mondo del lavoro, riescono già a pensare e ad agire in termini di salute e sicurezza. Questo perché siamo convinti che quello della sicurezza è essenzialmente un tema a valenza culturale. Occorre promuovere, iniziando dai giovani, una cultura della sicurezza. La nostra astensione, che speriamo possa essere modificata in Aula da quello che sarà l'atteggiamento della stessa Assemblea nei confronti degli emendamenti presentati, deriva essenzialmente dall'approccio al tema della sicurezza, approccio che traspare in tutto il disegno di legge; un approccio formalistico basato su regole e relative sanzioni e pene, che vengono in questo disegno di legge fortemente inasprite e che poi - come dimostra l'esperienza - rimangono sistematicamente sulla carta in attesa dell'immancabile condono. In materia di sicurezza - lo vogliamo ricordare all'Aula - il vero problema è l'effettiva applicazione delle norme, che può essere realisticamente affrontato solo mettendo da parte il tradizionale atteggiamento formalistico che tanto condiziona i comportamenti sui luoghi di lavoro. Che l'approccio del disegno di legge delega all'esame sia essenzialmente formalistico sanzionatorio lo dimostra il contenuto della lettera riguardante la riformulazione e la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale. Una legge delega che dovrebbe fissare solo i criteri e i princìpi si premura invece di indicare l'entità delle sanzioni incorrenti in una chiara violazione formale. Nel merito, il capitolo sanzioni presente nel disegno di legge delega è particolarmente gravoso, specialmente per le piccole e medie imprese. Combinando infatti il forte inasprimento delle sanzioni previste nello schema di legge delega con il già vigente appesantimento delle sanzioni introdotte in finanziaria si ottiene un grado eccessivo di pressione repressiva. Per questo motivo avremmo preferito una tecnica legislativa più per obiettivi che per regole, attraverso normative non solo più facilmente accessibili, ma - quel che più conta - adattabili ai diversi contesti organizzativi e alle modalità oggi sempre più differenziate e articolate di lavoro. A questo proposito, vorrei ricordare che da più parti, da sinistra e da destra (più da sinistra che da destra), si sostiene che l'incremento del fenomeno infortunistico è in larga parte addebitabile ai recenti cambiamenti che hanno interessato il mondo del lavoro e della produzione e i contesti organizzativi. Si dice che il ricorso alle esternalizzazioni, il ricorso eccessivo ai subappalti e ai lavori atipici, la compresenza nei luoghi di lavoro di lavoratori con differenti regimi legali e contrattuali sia causa di un aumento sia causa di un aumento del tasso di incidenti sui luoghi di lavoro. Se questo è vero - e d'altra parte riteniamo improponibile e impraticabile il ritorno ai vecchi modelli produttivi e lavoralistici del passato - è anche vero che questo fenomeno non si può combattere con un inasprimento delle sanzioni (che nulla hanno a che fare con la logica promozionale e preventiva); e non si può combattere con il formalismo, che mal si combina con i nuovi contesti produttivi e organizzativi. Formalismo e sanzioni eccessive, anzi, possono disincentivare le imprese (specie quelle piccole e medie) a ricercare modelli organizzativi moderni che rendano effettivo il rispetto della sicurezza. A questo proposito andrebbero valorizzate (ciò che il disegno di legge non fa in maniera compiuta) le norme di buona tecnica e di buona prassi

così come non vengono valorizzati dal disegno di legge delega gli organismi bilaterali, che oltre a poter svolgere un ruolo fondamentale nell'organizzazione dei modelli produttivi ai fini della sicurezza, oltre a poter svolgere una funzione appropriata per quel che riguarda la formazione e l'informazione, per il fatto stesso di avere al proprio interno lavoratori e datori di lavoro potrebbero svolgere una sorta di controllo sociale.

affronta uno tra i temi più scottanti posti all'attenzione dell'opinione pubblica negli ultimi tempi. Si tratta sostanzialmente della delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. La questione della sicurezza sui luoghi di lavoro è esplosa all'indomani di una sostanziale *escalation* di infortuni, che ha visto tagliare trasversalmente tutto il nostro Paese, tant'è che se oggi c'è un dato che accomuna è che il problema viene sofferto non solamente nel Meridione d'Italia ma anche molto al Centro-Nord, a dimostrazione dell'assoluta necessità di individuare i motivi di questo fenomeno e quindi di analizzare gli strumenti più importanti e più idonei per poterlo contrastare adeguatamente. *escalation* ha fatto sì che si aprisse un momento di confronto, di dialettica molto interessante, di prese di posizione di autorevoli comparti istituzionali del nostro Stato, ad iniziare dal Presidente della Repubblica, ma ha mosso anche le più alte gerarchie religiose. Diventa infatti estremamente difficile, negli anni 2000, dover assistere impotenti, giorno dopo giorno, ad uno stillicidio di vite umane senza che il legislatore possa far nulla per contrastare, ridimensionare, eliminare il fenomeno. C'è un dato

oggi impone una riflessione soprattutto se si guarda con attenzione alla caratteristica della più alta percentuale delle vittime. Si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di giovani molte volte assunti da pochi giorni, alle prime esperienze di lavoro, il che dovrebbe imporci un'adeguata riflessione sulla necessità di dare vita ad una nuova forma della cultura della sicurezza e anche ad una nuova forma di professionalizzazione, elemento senza il quale probabilmente nessuna normativa può determinare le condizioni per produrre efficacemente i suoi effetti.

Tutto va bene, quindi, quando si parla di riordino e di riassetto e quando si ritiene assolutamente doveroso ed opportuno inserire all'interno di un testo unico tutta la normativa, in modo da semplificarla, razionalizzarla, renderla più intelligibile. Ma, semmai, vi è un contrasto stridente con il provvedimento che oggi è sotto gli occhi di questo ramo del Parlamento: il fatto che con la procedura della legge delega, i tempi si allungano notevolmente fino a quando il provvedimento medesimo potrà produrre i suoi effetti, mentre in Italia si vive oggi una emergenza, sotto questo profilo, che avrebbe avuto bisogno di altri strumenti e di altre metodologie. Lo diciamo ovviamente con spirito molto costruttivo, nella consapevolezza che tutte le parti politiche debbono contribuire al miglioramento di un testo, sul quale evidentemente avremo occasione di esprimere le nostre valutazioni. Credo, però, che sia importante all'interno di questo provvedimento lasciare uno spazio significativo alla verifica del livello di applicazione della normativa esistente e dei motivi per i quali la stessa è stata larghissimamente disattesa e disapplicata. ne è un esempio plastico: è sotto gli occhi di tutti che esso non è stata applicato non solo dalle piccole imprese, cioè da quelle che non hanno le risorse adeguate per poter sostenere i costi di una riforma che andava impostata in una certa maniera, no; se andiamo anche all'interno dei cosiddetti enti pubblici, molti di questi dovrebbero chiudere le loro strutture per una violazione aperta dei princìpi e dei dettati Il problema è che le norme non si costruiscono a tavolino, ma bisogna calarsi nella realtà italiana, comprenderla, analizzarla e, quindi, produrre momenti di sintesi politica e legislativa. E per fornire un contributo - spero puntuale - alla valutazione, siccome la stragrande maggioranza degli infortuni sul lavoro, compresi quelli mortali e quelli che danno luogo ad invalidità permanenti, avvengono nel cosiddetto sistema di imprese, non può sfuggire al Parlamento il dato che il sistema di imprese in Italia oggi è diviso in tre fasce. Vi sono le imprese che non applicano *in toto* il contratto collettivo nazionale di lavoro: esse rappresentano un segmento significativo che, a mio personale avviso, va perseguito perché queste cosiddette imprese vanno assolutamente espulse dal mercato, creando all'interno dello stesso una distonia capace di produrre effetti devastanti. è un altro tipo di impresa che, invece, rispetta in maniera puntuale i contratti collettivi nazionali di lavoro. Lo può fare perché magari ha un'organizzazione storica alle spalle; perché ha una solidità economica collaudata; perché anche l'imprenditore stesso ha una cultura del fare impresa che si concilia e coincide sicuramente con il cosiddetto dettato costituzionale. poi un terzo segmento di impresa, il più ampio a mio avviso, costituito da quelle imprese che non operano pienamente nella cosiddetta legalità, non applicano cioè completamente i contratti collettivi nazionali di lavoro, ma vi si avvicinano molto.

Credo che su queste imprese, per esempio, bisogna fare una riflessione per aiutarle a rientrare in un sistema di piena legalità, creando quindi le condizioni ed i presupposti di base perché, insieme al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, insieme all'adempimento degli oneri previdenziali, della imposizione fiscale, vi sia anche l'adempimento sulle materie relative alla sicurezza sul lavoro. Oggi però non possiamo fare a meno di osservare quanto è sotto i nostri occhi. I problemi nell'ambito della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro sotto l'aspetto personale e umano del lavoratore nascono da una scarsa qualificazione professionale derivante da molti fattori. Molte volte c'è scarsa propensione alla propria qualificazione e riqualificazione professionale, ma altre volte c'è l'indisponibilità dell'impresa a determinare tali condizioni. Bisogna affrontare gli aspetti negativi per emarginarli o marginalizzarli e saldare invece gli aspetti positivi che si possono riscontrare su entrambi i fronti, perché sia superato questo *handicap* di natura culturale. Il secondo motivo deriva dalla cosiddetta eccessiva mobilità delle funzioni. Il personale scarsamente qualificato è disponibile a fare qualsiasi tipo di lavoro, anche con funzioni completamente diverse, diametralmente opposte, incapace quindi di poter garantire una perizia, un'esperienza, una competenza specifica anche per quanto riguarda le attenzioni che lo stesso lavoratore deve porre in essere sul tema della sicurezza del lavoro. Il terzo punto è legato alla precarietà contrattuale.

sia pure specifica, senza rimuovere le cosiddette situazioni di contesto non riusciremo sicuramente a raggiungere tale risultato. Né si può pensare che la risposta che possiamo dare e quindi il risultato che possiamo ottenere sia strettamente o direttamente collegato all'entità delle sanzioni che di fatto vengono applicate: non può essere solamente questo. Ci deve essere sicuramente anche questo: un impianto sanzionatorio serio che crei effettivamente le condizioni per aggredire il patrimonio del titolare dell'impresa che non rispetta le disposizioni di legge; però, per rendere efficace anche questa norma, le sanzioni debbono essere eque, quindi non debbono essere talmente basse da poter essere giudicate risibili, né talmente alte da determinare contenziosi lunghissimi sui quali poi si innestano procedure che sfuggono al principio di effettività.

effettuare una verifica sul campo. Non vengono rispettati i contratti collettivi nazionali di lavoro e, insieme con questi, non vengono rispettate neanche le condizioni della sicurezza; è un fatto oggettivo legato all'effettivo costo e all'effettiva

quelle che cioè operano all'interno di un sistema previdenziale, assistenziale e antinfortunistico riconosciuto. Molto spesso, gli organismi di controllo si premurano di effettuare delle verifiche proprio su queste, tralasciando invece l'area del lavoro completamente in nero e completamente sommerso, che in molti casi si può determinare attraverso l'ausilio e l'utilizzo di manodopera clandestina.

prevenzione, vigilanza ed eventuale repressione. Nella passata legislatura, insieme con il presidente Tofani, ho avuto la possibilità di effettuare verifiche in molte parti

riduce a 300 unità il numero di potenziali nuovi ispettori, mentre nel testo elaborato dalla Commissione,

Quindi, la penuria di soggetti utilizzati in azione di prevenzione, vigilanza e repressione di illeciti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è un problema importante, senza risolvere il quale non è possibile fare alcunché,

in caso di infortuni sul lavoro, non possono essere destinatarie di addebiti di natura colposa, ma di addebiti di natura dolosa. Mi riferisco al fenomeno delle cosiddette aziende madri che subappaltano ad aziende fantasma fasi di lavorazione estremamente difficili, pericolose e molto impegnative. traslano, sostanzialmente, su aziende fantasma le responsabilità patrimoniali, civili e penali derivanti da un'inosservanza della normativa in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro.

sotto quello sociale. Essi diventano, sostanzialmente, irresponsabili nei confronti delle rivendicazioni dei soggetti che dovessero attentare o aggredire il patrimonio

ma anche per il merito della materia, c'è bisogno di definizioni precise sulla efficacia del provvedimento stesso. Avere focalizzato l'attenzione della delega soprattutto sull'aspetto sanzionatorio,

alle proposte, alle direttive, alle iniziative che si dovranno adottare in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, il Governo sia disponibile a recepire questi indirizzi.

viene rilevata sostanzialmente non solo dalla qualità della vita media ma anche dalle condizioni di sicurezza e di salvaguardia di coloro che, più esposti di altri a fenomeni pericolosissimi per la loro salute ed integrità, debbono essere tutelati nella maniera migliore possibile. Spero quindi che il provvedimento in esame possa incontrare un decorso positivo

Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, ritengo, signor Sottosegretario, che questa mattina avrebbe dovuto farle compagnia un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico perché questa iniziativa, certamente lodevole, del riordino della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro va nella direzione di mettere ordine in un groviglio di norme che vengono da lontano e che hanno accompagnato ed assistito il divenire socio-economico di un Paese che, prendendo le mosse da una realtà oltremodo dilaniata quale quella che usciva dalla guerra negli anni '50, è pervenuto al rango di quinta potenza industrializzata del mondo. Attraverso la lettura di queste norme via via stratificatesi si legge evidentemente la storia economica di un Paese che cresce, la cui legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro è correlata strettamente al prodotto interno lordo e alla capacità di un popolo di crescere e di svilupparsi. Per essere chiaro, ritengo che la legislazione che oggi intendiamo darci con il costruendo testo unico non poteva certamente essere né desiderata né costruita né applicata negli anni '50, come non potrebbe essere applicata in Stati che non abbiano conseguito il livello di sviluppo di questo nostro amato Paese. Pertanto, prima ancora di pensare alle sanzioni e nella consapevolezza che quelle più rigorose non rimuovono mai le caratteristiche di base di un Paese che merita di essere vestito anche da un punto di vista giuridico e sanzionatorio, per quando e se si violano le norme, ritengo sarebbe stato più opportuno presentare innanzitutto un provvedimento con il quale si postulasse uno sviluppo economico ulteriore nelle aree laddove

Non giovò ad alcunché, non si riuscì a rimuovere quella pratica non virtuosa di produzione in frode. La sanzione pesante, quindi, non risolve il problema

Si vada pure nella direzione di mettere ordine, ma avremmo fatto soltanto un'esercitazione di costruzione di norme giuridiche se non pensassimo innanzitutto a leggi e a soluzioni che consentano di modificare l'indice di disoccupazione nelle aree laddove l'impresa in quanto tale non esiste ma è soltanto un'iniziativa di qualcuno che, per poter sopravvivere, pensa di realizzare un insieme di uomini e mezzi per produrre al peggio servizi e beni, senza soddisfare l'esigenza primaria di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. E allora, con questa convinzione, nella certezza che forse si perverrà pure alla costruzione di un testo unico, ma che esso non risolverà il problema al quale è diretto, mi rivolgo a lei, signor Sottosegretario: dica al Ministro dello sviluppo economico assente che, fin quando non ci saranno le condizioni ideali perché un'impresa possa produrre reddito e fin quando ci sarà un Governo che perseguita l'imprenditore per operare un prelievo fiscale sempre più sostenuto, aumenteranno forse le entrate e ci saranno pure i «tesoretti», ma certamente aumenterà la violazione delle norme in materia di tutela di salute e di sicurezza sul lavoro. Per tali motivi Forza Italia si astiene dal voto su questo provvedimento.

In Europa si registrano 4,5 milioni di infortuni annui, 4.600 dei quali mortali. In Italia è nota la situazione: 1 milione di infortuni l'anno, 1.302 mortali nel 2006. Vorrei qui ricordare il giovane Andrea, che è morto ieri dopo giorni di coma. coma. Lavorava in un'azienda dell'appalto dell'ILVA di Taranto, di quello che resta della nostra siderurgia. Nel 2006 sono morti 1.200 uomini e 101 donne sul lavoro.

all'interno di quel contesto. Hanno cioè riproposto al Paese, con un'iniziativa forte, una critica alle condizioni del lavoro e alla flessibilità e alla precarietà del lavoro. Ritengo sia stata un'iniziativa importante, forse bisognava dare più continuità, ma che ha contribuito senz'altro alla crescita di un senso comune sui temi della salute sul lavoro.

anticipano anche i contenuti del provvedimento che stiamo discutendo. Eppure il nostro Paese ha avuto una cultura forte, quella che si è chiamata il modello operaio di tutela della salute nei luoghi di lavoro. È sufficiente qui ricordare le dispense della Federazione lavoratori ma i processi di ristrutturazione delle imprese in questi anni hanno contribuito a rendere più precaria e più difficile quella condizione di lavoro, perché gli incidenti che prima ricordavo, che sono costanti nel tempo, accadono con una riduzione delle ore lavorate in particolare nei settori più colpiti dagli infortuni.

alto punto del rapporto tra democrazia e capitalismo, tra Stato e mercato e la controffensiva capitalista.

l'Assemblea di Confindustria, dove si è proposta una competizione tra l'*élite* capitalista, il sistema politico ed uno degli elementi che in tutti i Paesi del mondo, in particolare in quelli sviluppati, accompagnano i fenomeni della globalizzazione, vale a dire lo spostamento di decisioni strategiche dall'area democratica a quella capitalista

Siamo in presenza (va anche detto, perché non tutto il sistema delle imprese è uguale) di un conflitto tra i travolgenti predatori, come sono stati chiamati, in cerca di rapidi guadagni e invece una imprenditoria innovatrice, capace

anche le modalità con cui ragioniamo sul nostro PIL, sul prodotto interno lordo, dentro al quale sono ricomprese le rendite dell'INAIL per infortuni gravi e mortali.

corso alla riforma sanitaria, separando l'INAIL che assicura i lavoratori dal riconoscimento delle malattie professionali, che andrebbe invece assegnato alle aziende sanitarie.

incidenti e le morti sul lavoro sono appunto una lordura interna prodotta non da casualità. Ho epurato dai dati

della struttura produttiva e di situazioni produttive particolarmente nocive e disagiate e di effetti che si producono in termini di infortuni e malattie professionali sui procedimenti tecnologici e sulle sostanze usate; e c'è una diffusa disapplicazione della legge, nei fatti l'impunità per i datori di lavoro.

70 unità dei vigili del fuoco - cui va riconosciuta una capacità una professionalità di intervento alta - e 21 mezzi di spegnimento. La relazione dei Vigili del fuoco afferma che quanto si è manifestato era al di sopra di ogni previsione; diversamente dal ritrovarsi ad affrontare un evento in ambito petrolchimico, dove l'allarme sarebbe stato colto immediatamente dagli addetti ai lavori,

e che invece, stante la diversa struttura produttiva nel nostro Paese, è profondamente presente. Mi riferisco al lavoro domestico professionale, di quello obbligatoriamente iscritto all'INPS.

stati 2.767, di cui 2473 a donne. Qui, sì, c'è una condizione di genere nel lavoro da affrontare che la legge delega non fa in maniera prescrittiva, ma su cui è in necessario, invece, ragionare e intervenire a tutela della salute e della condizione della sicurezza. Ritengo che si stia consegnando alla discussione dell'Aula un provvedimento che consente una possibilità di intervento in più, anche prefigurando nuove figure di lavoratori responsabili per la sicurezza, come quelli di sito, assumendo, da questo punto di vista, anche accordi sindacali, come avvenuto per la costruzione della centrale di Civitavecchia, che hanno previsto il rappresentante della sicurezza indipendentemente dalle aziende che nel cantiere lavorano. Penso però

nella formula del *general contractor* è consentito il ribasso anche sulla quantità di denaro previsto per le norme di sicurezza.

- nella legge sono contenute anche norme per il contrasto al lavoro nero - ad una ricomposizione dei cicli produttivi e ad una qualificazione della nostra impresa. È pure un problema di dimensione dell'impresa

contro gli infortuni e le morti sul lavoro.

di avere un responsabile per la sicurezza, non hanno un *team* che lavori per mettere in sicurezza l'azienda. Credo che questi siano i reali motivi per i quali la maggior parte degli incidenti si consuma all'interno delle piccole aziende.

c'è un eccesso di sanzioni e di burocrazia; non vengono individuati all'interno dell'apparato produttivo le reali divisioni tra grande azienda, piccola azienda e lavoratori autonomi; i contenuti

con la semplificazione con la quale abbiamo approcciato quel testo unico, con l'armonizzazione di tutte le leggi vigenti che in qualche modo si sono incastrate all'interno di un quadro di riferimento

di una legislazione per la sicurezza che deve fare incentivazione, deve stimolare le imprese a produrre in sicurezza e deve fare cultura per la sicurezza. Non vedo e non ho colto, all'interno di questo provvedimento, la volontà di intervenire sugli appalti, che tutti dicono sia impossibile che continuino ad essere solo al massimo ribasso; non vedo tuttavia attività premianti in appalti che possano, appunto, premiare chi predilige il fenomeno della sicurezza nei cantieri. Uno scenario nuovo, assolutamente diverso, che ormai muta costantemente, e una dinamica del mondo del lavoro che non ci mette nelle condizioni di fotografare in maniera ferma questo fenomeno (penso all'*outsourcing*, al decentramento produttivo e a una serie di diversità rispetto al passato) ci impongono di vedere la materia in maniera snella, semplificata ed incisiva. Questo non è stato fatto e non sarà fatto dal Governo. Per di più, dopo un primo probabile tentativo di propaganda rispetto alla materia affrontata, vedremo scorrere davanti a noi mesi e mesi nei quali puntualmente i giornali e i telegiornali riporteranno

che, a detta di loro stessi, è così importante ed urgente. Non è così che si risponde ai problemi del Paese, non è così che si contribuisce a modernizzare il Paese e il suo apparato produttivo; non è questa la risposta che si aspettavano gli italiani.

Presidente, si apprende da una notizia di agenzia che sarebbe stata rinviata la cerimonia relativa all'insediamento del nuovo Comandante generale della Guardia di finanza,

Apprendiamo questa notizia su un evento che noi avevamo contestato, ieri ed oggi, anche con interventi in Aula di colleghi dell'opposizione, lamentando un ulteriore strappo alle regole che si stava per consumare: l'insediamento di un nuovo Comandante generale in assenza di un provvedimento di approvazione da parte dell'organo di controllo, la Corte dei conti, che notoriamente aveva chiesto chiarimenti al Governo sulla legittimità dell'articolazione dell'atto di nomina del nuovo comandante in assenza della precedente revoca. Avevamo lamentato questo strappo;

di invitare al più presto il Governo a riferire sulle motivazioni che lo hanno portato a questa scelta e sullo stato complessivo dell'*iter* procedurale relativo alla legittimità o meno

sconcertato di fronte a quanto sta succedendo e a poche ore dalle manifestazioni nei *no global* in occasione della visita del presidente Bush, e quindi alle solite devastazioni

proclamandosi difensore dei poveri e poi alla fine fa assistere la popolazione ad immagini sconcertanti di gente che commette reati di fronte alle telecamere nella più assoluta impunità

le chiedo anche di farsi parte diligente presso il presidente Marini affinché convochi al più presto una Conferenza dei Capigruppo per definire un calendario certo. Siamo in una situazione che credo non si è mai verificata nel nostro Paese sino ad oggi, se non in tempi bui di alcuni generali - quelli sì veramente infedeli - di tempi passati.

Presidente, credo che la notizia data dal collega Schifani e riportata da una agenzia di stampa possa essere immediatamente commentata da un rappresentante del Governo.

il vecchio Comandante della Guardia di finanza, che ha salutato i suoi uomini, ha ricevuto un applauso di cinque minuti, cosa mai avvenuta nella storia delle consegne tra comandante e comandante. Quindi, abbiamo di

questa mattina ha chiesto per prudenza, in attesa della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto di nomina, di sospendere

Se il motivo fosse che il Presidente del Senato è intervenuto, magari in ossequio alla richiesta dell'opposizione per ottenere questo risultato, le proteste per un risultato ottenuto grazie agli interventi di questa mattina francamente sarebbero un nonsenso. Signor Presidente, aprire una discussione

Signor Presidente, intervengo a nome dell'UDC per sollecitare la richiesta che ha avanzato il senatore Schifani. Schifani. Non trovo banale o superfluo discutere di questo argomento perché ci troviamo di fronte ad un fatto gravissimo, che è ancor più grave se il Governo ha rinviato la sua decisione a seguito della richiesta avanzata oggi in Aula.

finestra"). A titolo di informazione rispetto alla precedente agenzia, se ne è aggiunta un'altra che confermerebbe da parte dell'Ansa questa tesi; visto, però, che il Presidente è stato incaricato di dare questa risposta, credo che una risposta

e poiché non intendiamo assolutamente porre in essere qualsiasi forma di speculazione politica su un atto così grave qualora venisse confermato (del resto lei,

Certo, Presidente. Non è sulla stessa questione. Del resto, ho troppo rispetto per lei e per il presidente Schifani per potermi ripetere su considerazioni già fatte ed in maniera assolutamente esauriente. Vorrei segnalare a lei, signor Presidente, e ai colleghi, che da notizie di agenzia riportate peraltro già da qualche quotidiano nella giornata odierna, ieri si è verificato un fatto estremamente grave nell'ambito del Consiglio dei ministri dell'agricoltura, riunito a Lussemburgo. È stata infatti elevata

in minoranza e non è riuscito a conservare una minoranza di blocco, servita prima per sventare questa minaccia che mette a repentaglio l'esistenza stessa di decine di migliaia di aziende agricole italiane e getta anche nella confusione più totale milioni di consumatori. nostra impressione è che il Governo non abbia avuto una posizione concertata al proprio interno. Abbiamo l'impressione, anche leggendo le agenzie, che tra il Ministro dell'agricoltura ed il Ministro dell'ambiente vi siano posizioni molto diverse; abbiamo la certezza che la più grande organizzazione agricola italiana, la Coldiretti, ha attaccato pesantemente il ministro De Castro, accusandolo di non essere stato chiaro nella gestione di questa problematica così rilevante e delicata in sede comunitaria. Chiedo

all'Aula in ordine alla conclusione, assolutamente negativa per noi, di questa trattativa a Bruxelles. Tra l'altro, mi sembra che la minoranza di blocco sia venuta meno in quanto la Polonia si sarebbe sfilata in cambio di vantaggi - da essa ottenuti, non dall'Italia - nell'ambito della riforma dell'Organizzazione comune di mercato del settore degli ortofrutticoli, altro settore importantissimo. Abbiamo l'impressione, signor Presidente, che il Governo le stia prendendo di santa ragione a Bruxelles. Vorremmo quindi avere informazioni al più presto dal ministro De Castro. Colleghi, ritenendo sia ormai invalsa l'abitudine, per me disdicevole, per la quale ogni tanto qualcuno si alza e interviene sull'ordine dei lavori utilizzando tale sistema come strumento per parlare di qualunque tipo di argomento, il che non credo sia previsto dal nostro Regolamento (questi non sono,

finalizzato al riordino della disciplina in oggetto; esso è finalizzato a superare le cause degli inaccettabili incidenti nei luoghi di lavoro, ponendosi in linea con il recente richiamo del Presidente della Repubblica circa l'esigenza di assicurare un'effettiva tutela e sicurezza e con l'allarme delle organizzazioni sindacali; i numerosi incidenti sono favoriti - fra l'altro - dalla scarsa disponibilità di mezzi delle amministrazioni deputate al controllo del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché da meccanismi di attribuzione degli appalti che tendono a favorire le imprese meno scrupolose e, in generale, una scarsa chiarezza rispetto all'individuazione delle responsabilità; espresso apprezzamento per i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, ed in particolare per i seguenti: la valorizzazione degli accordi aziendali e, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi, al fine di orientare i comportamenti dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, verso il miglioramento dei livelli di tutela; la definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, attraverso: l'adozione di meccanismi di definizione, mediante il concorso delle pubbliche amministrazioni e delle parti sociali, di progetti formativi; il finanziamento da parte dell'INAIL degli investimenti in materia di salute e sicurezza su lavoro delle piccole e medie imprese; la promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei princìpi di autonomia didattica e finanziaria; la razionalizzazione ed il coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza al fine di rendere più efficaci gli interventi di programmazione, promozione della salute e vigilanza; il miglioramento dell'efficacia della responsabilità solidale tra committente ed appaltatore, nonché il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti. Essa fa riferimento anche all'adozione di meccanismi che consentano valutare l'idoneità tecnico professionale delle imprese e all'introduzione di condizioni di rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza sul lavoro ai fini sia della partecipazione alle gare di appalto e subappalto pubblici sia dell'accesso ad agevolazioni e finanziamenti a carico della finanza pubblica; la modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione stessa non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tali previsioni sono da accogliere con favore in quanto tese a garantire maggiore rigore in un settore nel quale la stessa competizione tra le imprese rischia di essere falsata a vantaggio dei soggetti in grado di ridurre notevolmente i costi sacrificando la sicurezza dei lavoratori; la revisione delle modalità di attuazione dell'eventuale regime di sorveglianza sanitaria, adeguandolo alle caratteristiche organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazione ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia; l'impossibilità che i decreti legislativi possano disporre un abbassamento dei livelli di sicurezza e di tutela o una riduzione delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze; preso altresì atto delle disposizioni in materia di sanzioni penali ed amministrative, relative alle violazioni delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute nel luogo di lavoro, di cui sarebbe opportuno valutare un ulteriore inasprimento rispetto ai casi di omicidio colposo e lesioni colpose; colpose; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni: 1) appare necessario che il disegno di legge assicuri l'adozione in tempi brevi di forme di coordinamento, a livello nazionale e territoriale, delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Queste forme di sinergia, infatti, consentono di sopperire, benché solo parzialmente, alle carenze di organico o di risorse finanziarie, che attualmente presentano le amministrazioni pubbliche competenti nel settore della sicurezza; 2) l'implementazione delle forme di coordinamento, tuttavia, deve essere accompagnato da un potenziamento, anche quantitativo, delle medesime amministrazioni pubbliche, al fine di elevare il livello di attività di prevenzione e di vigilanza; 3) con specifico riguardo alle aziende sanitarie locali (ASL), si rileva l'esigenza della definizione di un limite minimo di risorse finanziarie da destinare alla prevenzione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; tale valore potrebbe essere determinato in una percentuale del complesso della spesa sanitaria corrente delle ASL, ferma restando, in ogni caso, l'attribuzione di livelli quantitativi adeguati. Sarebbe poi opportuno che i proventi derivanti dall'attività di vigilanza delle ASL siano destinati all'attività di prevenzione delle stesse (attualmente, le regioni presentano un quadro eterogeneo riguardo l'impiego di tali risorse); appare opportuna l'istituzione di un libretto sanitario in cui si indichino (fermo restando il rispetto del diritto alla riservatezza) i fattori a cui il lavoratore sia esposto, ovvero sia stato esposto in precedenti attività, e che potrebbero determinare l'insorgenza di una malattia; 5) occorre, inoltre, sia assicurare il pieno funzionamento degli attuali sistemi di "registrazione" di malattie professionali, come quelli relativi ai tumori ed ai casi di asbestosi e di mesotelioma asbesto correlati, sia estendere i medesimi sistemi ad altre malattie; 6) si invita a riporre attenzione all'esigenza di garantire efficaci forme di tutela nei confronti delle donne lavoratrici, anche in relazione alle specificità di genere; 7) si sollecita una particolare attenzione nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori domestici, ai quali occorre, in prospettiva, assicurare idonee forme di tutela; 8) con riferimento alle figure professionali del sistema di prevenzione aziendale di cui all'articolo 1, comma una, lettera *g)*, si segnala l'opportunità di tenere conto delle disposizioni attualmente in vigore. Con particolare riguardo al potenziamento delle funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, si tratta di questione che è auspicabile affrontare attraverso il coinvolgimento delle parti sociali; 9) relativamente ai soggetti che partecipano, a vario titolo, al sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *n)*, si valuti l'inserimento anche dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e delle università; 10) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera *s)*, in materia di rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, si consideri l'opportunità di una più articolata definizione dei principi e criteri con cui la delega legislativa deve essere esercitata; esercitata; 11) si sollecita un incremento delle risorse finanziarie da destinare alla tutela della salute dei lavoratori, ai sensi del decreto legislativo n. 626 del 1994». Nel ringraziare tutti i componenti della Commissione che hanno sottoscritto e condiviso il parere da me esteso ed anche la Presidenza che ha permesso di porre questo importante parere all'attenzione dell'Aula,

sviluppò un antagonismo molto forte e rigoroso nelle Commissioni parlamentari e, nello stesso tempo, la Conferenza Stato-Regioni

Perché si sviluppò questa opposizione così dura? Dopo tutto questa è materia che avrebbe potuto dare luogo ad un atteggiamento *bipartisan* da parte degli schieramenti politici. La sinistra però in quell'occasione capì che il disegno di legge presentato dal centro-destra si ispirava soprattutto a criteri generali che non potevano essere condivisi non solo dalla sinistra radicale ma anche dalle cosiddette forze riformiste dell'allora opposizione. Il disegno di legge presentato dal Governo Berlusconi, infatti, faceva perno soprattutto sulle forme di controllo preventivo che, anzi, venivano definite forme di controllo sociale. cioè a definire un'azione di prevenzione diffusa sul territorio e capillare.

nel momento in cui un lavoratore ha la sfortuna di prestare la sua opera in un'azienda nella quale si incorre in determinate procedure,

della diversa posizione dei due schieramenti. Non è che noi non condividiamo questo provvedimento (siamo anzi stati promotori nella precedente legislatura, trovando voi fieri oppositori, di un disegno di legge sulla materia), ma siamo profondamente diversi per quanto riguarda poi l'approccio generale e la fase di razionalizzazione

paletti di verità perché fino ad ora sono state dette molte cose, ma le verità non sono emerse. Qual è la verità?

perché la sinistra, e non solo quella antagonista, ha sempre affermato che gli infortuni sul lavoro subivano un incremento in presenza di contratti di lavoro atipici; sosteneva la contrattazione atipica - sostanzialmente ciò che viene definito da quello schieramento come il diffondersi del precariato - provocava un incremento degli infortuni sul lavoro. Invece no, invece proprio la cosiddetta

gli infortuni sul lavoro sono aumentati? Perché c'è un nuovo processo di immersione di unità produttive e di lavoro. Questa è la verità. Se non prendiamo atto

non incrementare in maniera più che considerevole il numero degli ispettori sul lavoro? Perché non lo incrementate? Perché voi badate molto al momento sanzionatorio, signor sottosegretario Montagnino,

perché - guardate - con le sanzioni e le misure interdittive fino ad ora si è fatto ben poco. Dovreste piuttosto investire nella politica degli incentivi;

Le politiche di prevenzione si fanno anche con gli accordi con le associazioni di categoria, facendo in modo ‑ ad esempio - che, come si verifica già in molte aree della microimpresa dell'artigianato, quando si tra prestatore d'opera e imprenditore la si utilizzi? Perché non arrivare a queste forme d'intesa diffusa? Ecco allora che

chi poi utilizza in subappalto le imprese gestite avventurosamente e soprattutto

e di condivisione con una impresa a sfondo criminale, in cui l'imprenditore è sostanzialmente una figura criminale,

e incorre nelle sanzioni anche contro la sua volontà. Ricapitolando, non ci sono risorse per le politiche di professionalizzazione, non ci sono risorse per gli ispettori, esasperate gli adempimenti formalistici contro le piccole imprese, sanzioni che portano a misure interdittive radicali. Secondo me, questo disegno di legge non pone rimedio alle morti bianche e agli infortuni sul lavoro,

sanzioni durissime in genere c'è il sommerso e con questo tipo di norme rischiate di incoraggiare il sommerso. Avremmo

Signor Presidente, onorevoli senatori, signori del Governo, il ripetersi incessante di morti e infortuni sul lavoro ha costretto il Parlamento ad intervenire con urgenza in una materia, quale quella della sicurezza sul lavoro, da sempre all'attenzione dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e dell'opinione pubblica. L'alto, accorato ed autorevole richiamo del Presidente della Repubblica corrisponde al profondo sentire della nostra gente. Non possiamo più accettare che l'integrità della persona, la sua stessa vita, costituiscano una sorta di costo sociale. L'intento del Governo, con la proposizione del disegno di legge n. 1507, è certamente positivo. Sarebbe però molto ingenuo, e soprattutto fuorviante, anche solo ritenere che con questo nuovo provvedimento si risolveranno tutti i problemi della sicurezza sul lavoro, sia per ragioni di tempistica legislativa sia per ragioni contenutistiche. Un esame analitico delle disposizioni che vogliamo introdurre nell'ordinamento ci conduce a dire che la strada intrapresa è sicuramente quella giusta, ma con altrettanta tranquillità, o meglio preoccupazione, questo esame analitico mi consente di dire fin da ora che non sarà assolutamente sufficiente. La sicurezza sul lavoro è una questione dalle molteplici sfaccettature, che quindi deve essere affrontata sotto diversi punti di vista. È una questione di civiltà, una questione culturale, sociale, economica e di formazione. È un settore nel quale le fasi della prevenzione e della vigilanza assumono un ruolo rilevantissimo e nel quale ha un ruolo rilevante pure l'aspetto repressivo.

In materia di prevenzione, controllo e repressione, infatti, il mio giudizio sul disegno di legge è convintamente negativo. Osservo che due rimangono i punti critici fondamentali: la decisione politica di investire e di continuare ad investire in materia di prevenzione e vigilanza in mezzi, uomini e strutture in proporzione adeguata rispetto all'entità del fenomeno; la volontà politica del Governo, concreta, di far funzionare le strutture e i meccanismi di vigilanza, controllo e prevenzione. Non è, ovviamente, un problema soltanto del Governo, ma anche dei vari enti pubblici competenti in materia, a partire da Regioni e Province. Senza un impegno costante e pressante in tale ottica continueremo, purtroppo, a piangere lavoratori morti. A questi aspetti della sicurezza sul lavoro si collega strettamente tutta la tematica della repressione anche penale. In Commissione giustizia abbiamo espressamente affrontato la questione, dovendo esprimere un parere istituzionale sul disegno di legge n. 1507. La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprimeva un parere unanime contrario in materia di sanzioni. La Commissione inseriva altresì specifiche sollecitazioni ritenute qualificanti. Per quanto concerne il regime delle sanzioni, la Commissione riteneva che le soluzioni adottate fossero eccessivamente blande e non idonee a reprimere penalmente un fenomeno così grave. Perché dicevamo e continuiamo a dire questo? In particolare, l'indicazione delle sole sanzioni dell'arresto e dell'ammenda previste nei casi in cui le infrazioni ledano gli interessi generali dell'ordinamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per di più da comminare in via anche alternativa, risulta oltremodo effimera, perché configura le violazioni di norme antinfortunistiche da parte dei datori di lavoro o degli altri soggetti quali semplici contravvenzioni. Risulta inaccettabile, mentre continuano a verificarsi incidenti sul lavoro in ogni parte d'Italia, ogni giorno, e considerando la gravità sostanziale e sociale dei reati perpetrati, rispetto ai quali è palese la sproporzionata irrisorietà della sanzione penale proposta, e quindi la non dissuasività della medesima. Come è perfettamente comprensibile, l'entità microscopica della sanzione, la mortificante sproporzione tra la stessa e il titanico precetto del quale essa è posta a presidio rende desolantemente la norma proposta, come la stragrande maggioranza di quelle poste a difesa del lavoro e dei lavoratori, appena meno seria ed imperativa di una grida della Milano del XVII secolo. Inoltre, la scelta per la natura contravvenzionale delle sanzioni è tale da incidere pesantemente sul regime della prescrizione, considerando che i reati contravvenzionali si prescrivono in soli quattro anni. Questo costituisce un'amnistia costante. Alla luce di tali considerazioni, la Commissione riteneva unanimemente necessario procedere ad una correzione della parte relativa al regime delle sanzioni penali, prevedendo che i fatti più gravi, comportamenti, omissioni gravi in violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro dovessero essere puniti come delitti e quindi con la pena della reclusione e/o della multa e pertanto con termini di prescrizione sicuramente più elevati. A tal proposito, sarebbe auspicabile che il Governo o il relatore accogliesse la proposta unanime della Commissione giustizia e presentasse un emendamento specifico, quale quello che materialmente abbiamo già consegnato al relatore Alcuni degli altri punti qualificanti emersi sono i seguenti. Il primo attiene alla necessità di considerare adeguatamente il principio di precauzione (del quale non si fa cenno nel disegno di legge) come norma fondamentale e vincolante che ogni produttore, importatore, esportatore e/o commerciante deve applicare, ovvero deve documentare in modo rigoroso e preventivo alle autorità preposte l'innocuità a breve, a medio e a lungo termine della sostanza, del prodotto o della tecnologia che intende produrre, impiegare o commercializzare. A questo principio si collega la riconsiderazione di quanto sia pacifico, a livello scientifico, che non esiste un livello, una soglia o un limite che dir si voglia, per quanto infinitesimo, per le sostanze cancerogene e genotossiche al di sotto del quale non vi sia rischio oncogeno per le persone esposte e conseguentemente come tali sostanze debbano essere sostituite con quelle a dimostrata innocuità. Il riferimento è chiaramente a quanto avviene nel campo delle malattie professionali, ai danni ad esempio dei lavoratori esposti o ex esposti a sostanze cancerogene e genotossiche (come l'amianto o il cloruro di vinile monomero), che stanno pagando sulla propria pelle omissioni e manchevolezze da parte innanzitutto dello Stato. Né va taciuto il fatto che nel disegno di legge in questione non vi sia traccia dell'attivazione di una stringente normativa di prevenzione dei rischi lavorativi, con particolare riferimento - appunto - alle malattie professionali e agli infortuni, né vi sia cenno della dotazione al sistema prevenzionistico del Paese di appropriati mezzi (si intendono gli stanziamenti economici sul bilancio dello Stato); c'è, invece, un limitato e generico rinvio ad oneri sostenuti dall'INAIL nell'ambito della creazione di un organismo a base tripartita, peraltro in palese conflitto di interessi da parte dell'istituto assicuratore. cenno ad appropriati mezzi in dotazione al sistema prevenzionistico del Paese, al personale qualificato e alle strutture, ivi comprese quelle di ricerca a ciò finalizzate. Quanto alle altre parti del disegno di legge delega, alcune osservazioni devono essere svolte a proposito di temi non trattati o trattati in modo insoddisfacente nel provvedimento. La valutazione dei rischi dovrebbe riguardare, oltre quelli per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, anche i potenziali pericoli per la popolazione e per coloro che vivono attorno agli stabilimenti e ai siti industriali e commerciali di particolare rilievo, ma di ciò non c'è alcuna traccia né considerazione nel disegno di legge. Occorre inoltre introdurre misure di tutela più intensa per specifiche tipologie di lavoro, anche in considerazione della particolare nocività di alcuni ambienti di lavoro, compreso quello domestico, riservando altresì una specifica attenzione al lavoro precario e alla violenza psicologica. È necessario riconoscere poi concretamente il diritto, in capo alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei familiari delle vittime, di costituirsi parte civile nei procedimenti a carico del datore di lavoro per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. È opportuno predisporre idonee misure volte a garantire la gratuità del patrocinio legale alle vittime di incidenti sul lavoro e di malattie professionali e alle loro famiglie. Occorre regolamentare in modo più stringente la responsabilità solidale tra primo appaltatore e subappaltatori, introducendo l'obbligo giuridico di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali da parte del primo appaltatore nei confronti di tutti i subappaltatori successivi, confermando altresì l'obbligo di cooperazione e coordinamento tra committente ed appaltatore o subappaltatori, per prevenire i rischi derivanti dall'ambiente del committente e dall'interferenza tra i vari lavori. È necessario prevedere poi l'obbligo giuridico, per il datore di lavoro committente, di redigere un piano di sicurezza e di coordinamento che tenga conto dell'utilizzazione comune di infrastrutture, impianti e misure di protezione collettiva, nel quale siano definite anche le procedure da eseguire in caso di emergenza, le responsabilità del committente, il piano di sicurezza e coordinamento da allegare al contratto di appalto o di lavoro. Un ultimo punto concerne la necessità di creare un vero sistema di sorveglianza sanitaria, che riguardi anche gli ex lavoratori (cioè i lavoratori ex esposti o comunque coloro che sono usciti dal mondo del lavoro), adeguando la sorveglianza sanitaria alle diverse forme organizzative del lavoro, alle varie e differenti esposizioni a sostanze tossiche o nocive, nonché ai criteri e alle linee guida scientifiche più avanzate, prevedendo strutture, sistemi e meccanismi di sorveglianza sanitaria, soprattutto a livello locale. Dall'illustrazione, pur sintetica, che ho effettuato emergono in maniera evidente le criticità e tutte le perplessità che ho maturato sul sistema sicurezza sul lavoro che viene proposto. Al termine della passata legislatura la Commissione d'inchiesta del Senato sulle morti bianche aveva concluso i propri lavori redigendo e approvando una relazione finale molto dettagliata e approfondita, che soltanto in parte è stata trasfusa nelle linee generali del disegno di legge che ci troviamo oggi ad affrontare e che invece avrebbe meritato una maggiore considerazione. Non finisce certamente oggi o nei prossimi giorni il nostro impegno e il nostro lavoro; purtroppo saremo costretti a tornare sulla materia, perché costantemente norme e controlli dovranno essere aggiornati e adeguati. Peraltro - e mi avvio alla conclusione - pur proponendo di accogliere il suggerimento unanime della Commissione giustizia per quanto attiene alla parte sanzionatoria e nonostante i punti critici rilevati, ritengo che vada dato un giudizio, anche se parziale, sostanzialmente positivo al disegno di legge n. 1507, che si mette lungo una via obbligata di tutela del lavoro e del singolo lavoratore. È solo un piccolo passo limitato, ma comunque utile, che avrà bisogno di ulteriori aggiunte e integrazioni.

il lavoro svolto dalla Commissione speciale nella scorsa legislatura, che ci ha lasciato del materiale prezioso, solo in parte - come ricordava ancora il collega Casson - proposto nel provvedimento che stiamo discutendo. provvedimento è data dai dati drammatici degli ultimi anni, che confermano una dinamica estremamente negativa. Non ci troviamo di fronte a un miglioramento della situazione, ma, anzi, le cifre ufficiali parlano piuttosto di un aumento degli infortuni del 2,2 per il 2005 e il 2006. È da rilevare anche - come già credo qualcuno abbia fatto in questa sede - che sono le lavoratrici ad esserne colpite sempre di più; anche le lavoratrici, entrate nel mondo del lavoro sempre più numerose. Per quanto riguarda il settore edile, tradizionalmente al centro degli incidenti, purtroppo si conferma una crescita degli incidenti, anche mortali. La FILLEA ha calcolato, nel 2006, 258 omicidi bianchi, con un balzo del 35 per cento rispetto all'anno precedente. A metà di aprile di quest'anno contavamo già più di 300 morti, 8.000 invalidi e 300.000 infortuni gravi. È una inaccettabile sequenza di tragedie, non una tragica fatalità ma un fatto materiale e sociale concreto, una guerra interminabile contro il lavoro o per meglio dire - usando le parole di un dirigente della FIOM - la guerra della competitività contro il lavoro. Al costo delle vite umane è chiaro che si aggiunge poi il costo economico e sociale: l'INAIL stima 35 miliardi di euro questo costo, cui si aggiunge quello delle malattie professionali, di 6,8 miliardi. Inoltre, bisogna sempre tenere conto che il dato degli infortuni è calcolato molte volte al ribasso, perché contemporaneamente esiste una stima che valuta tra il 10 e il 20 per cento il numero degli incidenti occultati. Ci troviamo di fronte - e certe volte le cronache lo rivelano - ad episodi abbastanza agghiaccianti: incidenti spacciati per incidenti stradali o domestici; qualche volta addirittura si cerca di coprirli come fossero suicidi o risse; si registra poi persino il disumano fenomeno dell'abbandono dell'infortunato grave che operava senza essere iscritto sui libri paga. È chiaro che se tutto ciò pesa moltissimo l'enorme esercito di lavoratori precari e di lavoratori in nero. Al centro degli incidenti abbiamo sempre la conferma che c'è la violazione della normativa, non solo delle normative più recenti ma anche di quelle più vecchie, più consolidate, quelle che datano addirittura già dagli anni Cinquanta, e l'assenza o l'insufficienza di protezioni ed inadeguatezze strutturali. Questa è la principale causa di morte sul lavoro. Solo recentemente peraltro, per quanto riguarda i cantieri edili, cantieri edili, con la finanziaria si è cercato di porre ostacolo al vergognoso fenomeno degli infortuni del primo giorno di lavoro: circa 250 incidenti mortali che altro non sono che l'indicatore tragico del lavoro irregolare che emerge soltanto al momento dell'incidente. dell'incidente. Sottolineo anche il fatto che la concentrazione degli infortuni nei primissimi giorni di lavoro è particolarmente accentuata nelle microimprese. In questo contesto bisogna anche ricordare che i lavoratori migranti - per esempio - nei cantieri costituiscono ormai il 50 per cento della forza lavoro e pagano un tributo di sofferenze e di sangue superiore alla media.

che spesso erano proprio i lavoratori precari non radicati nel contesto aziendale e sindacale, e quindi di fatto meno tutelati e meno formati, ad essere impegnati nello svolgimento di attività nocive. Quindi, siamo tutti d'accordo che è necessaria una nuova normativa, un testo unico, tanto più che i modelli produttivi affermatisi negli ultimi anni, a partire dal fenomeno della terziarizzazione dell'impresa, della dispersione della produzione sul territorio e della precarietà e della stabilità del lavoro, richiedono normative nuove. Sono tutti aspetti che, per quanto riguarda la sicurezza, appartengono non più solo ad alcuni comparti produttivi o di categorie di lavoratrici e lavoratori, ma stanno diventando comuni a tanta parte dell'industria e dei servizi. Dal tema della organizzazione del lavoro alle nuove forme di rappresentanza possiamo generalizzare problematiche e proposte che vengono da esperienze pilota o da riflessioni di settori come l'edilizia e la cantieristica. Le stesse responsabilità dell'impresa madre nella terziarizzazione devono essere riviste e potenziate, come già molti hanno sottolineato, come va rafforzata e coordinata, e dove è possibile unificata, la presenza dei rappresentanti dei lavoratori. Abbiamo un esempio di fronte a noi: la lotta dei lavoratori del porto di Genova, che ha portato generalmente ad un accordo che garantisce ai rappresentanti dei lavoratori maggiori poteri di controllo e prevenzione, maggiore indipendenza rispetto alle imprese e quindi anche maggiore efficacia; ciò può costituire un punto di riferimento importante. Non solo sono state approvate nuove forme di collaborazione tra le diverse autorità addette al controllo e alla prevenzione, ma soprattutto è stato costituito un organismo dei lavoratori che può rappresentare e coordinare la complessità delle mansioni e delle aziende che operano sulle banchine dopo che i processi di privatizzazione avevano frantumato il ciclo produttivo. La Commissione lavoro, credo, nel discutere la proposta di legge delega del Governo ha fatto un buon lavoro, introducendo una serie di emendamenti migliorativi, rendendo più stringenti alcune normative, impegnando anche il Governo a reperire le risorse finanziarie necessarie ai nuovi compiti, che non erano previste nel disegno iniziale, e consegnando quindi all'Aula una proposta più precisa e avanzata. Voglio tuttavia sottolineare, come ha già fatto il senatore Casson, alcuni punti di debolezza che ancora persistono e che vorrei superati attraverso l'azione emendativa.

Credo che non sia stato ancora dato il ruolo e i relativi poteri che dovrebbero essere dati agli RLS. È proprio dall'esperienza concreta del loro lavoro che è emersa in questi anni la richiesta che essi siano dotati di maggior potere di intervento. Il testo proposto non soddisfa ancora questa esigenza; certo, la debolezza degli RLS è anche il risultato dell'indebolimento complessivo del movimento sindacale, ma solo un rafforzamento normativo e una maggiore tutela darebbero agli RLS una piena indipendenza e capacità di resistere ai ricatti a cui sono sottoposti. In terzo luogo, credo non siano tenuti ancora in adeguata considerazione alcuni problemi, come la valutazione dei rischi per la popolazione, un'adeguata quantificazione degli organi di vigilanza rapportati al contesto produttivo, oppure il principio di precauzione rispetto a sostanze tossiche di cui non sia accertato il principio di pericolosità.

settore dove assistiamo a una particolare situazione in cui coloro che dovrebbero essere controllati sono nello stesso tempo i controllori. Occorre quindi a questo proposito una radicale modifica del decreto ministeriale n. 284 del 2000. Tutti i lavoratori del Ministero della difesa devono essere tutelati come gli altri: i controlli, le verifiche e la vigilanza devono essere effettuati dagli appositi dipartimenti delle AUSL. Solo in particolari aree dove può esistere effettivamente il segreto militare può essere previsto un accesso parziale o nessun accesso. A questo proposito ho presentato sia degli emendamenti sia una mozione che invita il Governo a rivedere il citato decreto ministeriale Voglio svolgere infine alcune considerazioni, forse un po' più politiche, non specifiche, ma che credo abbiano un rapporto molto stretto con quanto discutiamo oggi.

che, certo, hanno avuto anche il merito di porre all'attenzione dell'opinione pubblica il problema e di sollecitare il Parlamento a discuterne; in questo senso hanno giocato un ruolo positivo. Ma ho trovato anche tanta ipocrisia nelle cose scritte.

contraddittori. Voglio dire che se le scelte economiche e le ideologie dominanti restassero quelle della costante pressione sul lavoro, della riduzione del costo del lavoro, della ricerca del massimo profitto e della concorrenza senza vincoli, i fenomeni infortunistici, da tutti denunciati, non farebbero che perpetuarsi. È contraddittorio parlare di sicurezza e poi, ogni giorno, chiedere maggiore competitività, maggiore flessibilità, maggiore precarietà, quando esiste una pressione costante ad andare oltre le regole, a ottenere il massimo, a mettere sotto torchio lavoratrici e lavoratori sempre in nome del profitto e per battere la concorrenza. Non può essere sottaciuto che, ogni giorno, lavoratrici e lavoratori sono sottoposti a un costante ricatto sul proprio posto di lavoro, e che sono costretti non solo a lavorare di più, ma anche a correre il rischio dell'infortunio o della malattia, per difendere il posto di lavoro. È l'organizzazione capitalistica stessa del lavoro che uccide e che fa ammalare. Qualcuno di quelli che qualche volta fanno i Soloni nei giornali o nelle televisioni è mai andato a parlare a lavoratori e lavoratrici dall'uscita di un turno della fabbrica, a guardare i loro volti, la loro fatica? Riesca mai ad immaginare quali siano i tempi di lavoro e lo *stress* dentro un *call center*? E non faccio altri esempi. Un giorno si parla delle morti bianche e il giorno dopo sullo stesso giornale viene lanciata una campagna contro gli assenteisti o sul fatto di quanto poco si lavori in Italia rispetto a quell'altro Paese del mondo. Fantastico! Così qualcuno ha anche il coraggio di proporre l'abolizione della conquista storica del pagamento dei primi tre giorni di malattia, e qualcun altro di affidare a enti privati i controlli sulla sicurezza che non possono che spettare a una struttura pubblica. Infine, qualsiasi battaglia contro gli infortuni rischia di essere vana se non si mette mano alle leggi sulla precarietà (3 milioni di lavoratori e lavoratrici coinvolti, a cui si aggiungono i 3,3 milioni di quelli in nero, come ha spiegato il ministro del lavoro, Damiano). Doveva essere, questa della lotta alla precarietà, una centralità del Governo; tutta la maggioranza ha difeso quest'obbiettivo in campagna elettorale. Ad oggi siamo al palo. Nulla è stato fatto per abrogare o superare - non importa quale verbo usare - la legge n. 30 del 2003, legge della precarietà totale che ha consentito lo sfondamento delle regole giuridiche del mercato del lavoro, concedendone una frammentazione parossistica da cui derivano appalti, subappalti e via via, esternalizzazioni anche da parte delle aziende «serie». Se non interveniamo con misure drastiche contro la precarietà per rimettere al centro il diritto del lavoro, rischiamo che anche il positivo provvedimento che stiamo discutendo e che speriamo di approvare oggi resti lettera morta e non produca il cambiamento invocato. In conclusione, se non ci sarà una nuova sensibilità politica sociale che produca una rivalutazione dei diritti dei lavoratori, un nuovo protagonismo del movimento sindacale e, quindi, anche dei rappresentanti della sicurezza, è difficile pensare che nei luoghi della produzione e dei servizi, nelle imprese, nella società in genere si affermino le condizioni di un'efficace prevenzione. Per questo condivido largamente anche

e permanente nella realtà dei fatti all'interno della società, sui luoghi di lavoro. Sì, deve essere reintrodotta la centralità dell'articolo 1 della Costituzione italiana: «L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro». Ed io aggiungo: deve essere fondata sulla sicurezza del lavoro.

una premessa per tutti: è compito di tutti salvaguardare anche in maniera legislativa il mondo del lavoro e dei lavoratori. Premesso questo, credo sia però interessante inserire dei dati, altrimenti parliamo senza numeri. Riprendo i dati INAIL, riguardante il confronto tra il 2005 e il 2004 chiaramente degli infortuni denunciati, perché sappiamo benissimo che molti infortuni rimangono oscuri. Ebbene, nel raffronto 2004-2005 non possiamo non notare un sostanzioso calo degli infortuni sul lavoro. Unico dato in crescita è quello degli infortuni *in itinere*, passati dagli 84.500 del 2004 agli 87.000 del 2005. perdita di vite umane è da attribuire a una significativa contrazione dei casi mortali avvenuti *in itinere*: pur aumentando il numero degli infortuni sono calate le morti, che nel 2005 scendono a 280 casi, rispetto ai 301 del 2004, ai 355 del 2003, ai 396 (che fu un picco) del 2002. Sicuramente ciò è da attribuire agli effetti delle disposizioni in materia di circolazione stradale, almeno credo che l'unico motivo di cambiamento sia la cosiddetta patente a punti, che entrò in vigore proprio nell'anno 2003.

della produzione. È indubbiamente probabile, tant'è che nell'ultimo periodo in cui la produzione sta ripartendo c'è stato un netto incremento degli infortuni sui lavori.

Dicevo che il segnale è prodotto da una ripresa produttiva dell'intero Paese, anche perché dove non c'è stato un incremento di produzione, cioè nell'agricoltura, si è registrato un ribasso degli infortuni dell'ordine del 2 Questa è una storica perdita di occupazione nel settore dell'agricoltura, che ormai è da anni in calo. Per quanto riguarda la frequenza infortunistica per Regione, mi dispiace dover intervenire da umbro, perché noto che al primo posto c'è purtroppo l'Umbria, una piccola Regione: 800.000 abitanti, 600.000 elettori. L'Umbria è caratterizzata da una forte presenza di piccole imprese, soprattutto a carattere artigianale, e probabilmente in queste c'è minor controllo sulla protezione e sull'infortunistica;

Il nostro Paese presenta per gli infortuni nel loro complesso valori ben al di sotto sia della media europea sia dei Paesi assimilabili al nostro per cultura, economia e *Welfare*, come Spagna, Francia e Germania.

Ritorno al problema degli incidenti mortali *in itinere*, che sono oltre il 30

a salvaguardare i lavoratori nel loro percorso *in itinere*, in uscita e in entrata dai posti di lavoro. In realtà, questo Governo solo ultimamente si sta accorgendo della carenza di infrastrutture.

Per il CENSIS sono circa 5 milioni. Probabilmente, sono dati difficili da analizzare. Se andiamo a valutare l'entità del lavoro irregolare nelle Regioni

La classifica regionale, in percentuale, del rapporto tra lavoratori completamente in nero sul totale dei lavoratori irregolari,

Su 1.628 aziende ispezionate, ben 856 sono risultati irregolari. Su 1.028 lavoratori irregolari

Su 163 cantieri ispezionati, ben 130 sono risultati irregolari.

nuove norme tese ad incidere fortemente, non con sanzioni più pesanti delle attuali e basta, ma con finanziamenti significativi nei confronti dei controllori. Occorreranno senz'altro norme più significative dal punto di vista sanzionatorio ma, sicuramente, non dal punto di vista repressivo.

l'INAIL, i Vigili del fuoco, le ASL, i Carabinieri, la Polizia di Stato, le Regioni per le loro competenze, la polizia municipale e la magistratura). Ebbene, tutti questi organi, preposti al controllo,

Crediamo che occorra che lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore - perché no? - comprendano cosa significhi sicurezza nel proprio lavoro.

artigiani, lavoratori devono riunirsi attorno ad un tavolo per migliorare le conoscenze sull'infortunistica. Solo in questo modo potremmo arrivare ad un risultato.

riesaminato perché, se non c'è sanzione giusta e coerente, evidentemente regna l'indifferenza nel mondo del lavoro; si preferisce pagare un'ammenda se questa costa molto meno della protezione dei propri lavoratori.